io chiederei che si specificasse che la preclusione della seconda parte è stata determinata dalla reiezione da parte del Senato di identico ordine del giorno G9, recante le stesse parole. parole. Deve essere chiaro che il Senato ha respinto l'apprezzamento per la Guardia di finanza: questo è ciò che è avvenuto ieri. Dunque, non solo è stato approvato il comportamento del Governo, ma è stata anche respinta una proposta di apprezzamento della Guardia di finanza. dico questo perché - e spero siano stati compiuti gli atti che il presidente Caprili aveva assicurato questa mattina, quando sono intervenuto - da stamani il principale telegiornale del servizio pubblico sta diffondendo una notizia falsa

l'operato del Governo ed esprimeva apprezzamento per la Guardia di finanza". Ora, anche il presidente della Commissione di vigilanza Landolfi è intervenuto pubblicamente sul tema; il presidente Caprili mi aveva fornito ampie assicurazioni che il Senato sarebbe intervenuto con una nota ufficiale.

Ieri, nelle concitate fasi del voto sull'ordine del giorno approvato, ho chiesto ripetutamente e in modo molto visibile la parola per un richiamo al Regolamento e non l'ho ottenuta. Sono certo che si è trattato di una svista e che il Presidente non si è accorto della mia richiesta, come forse non si è accorto della richiesta di parola del senatore Malan. Malan. Mi rendo conto di essere un senatore di prima legislatura e che in certe situazioni concitate l'attenzione del Presidente, giustamente, si rivolge ai Presidenti di Gruppo e a senatori più autorevoli, ma vorrei soltanto che si evitasse anche solo l'impressione che i diritti dei senatori *peones*, quale io sono, soprattutto di opposizione, possano anche essere minimamente conculcati.

non solo è stato sensibile nel dibattito di ieri, ma lo è di norma, anche guardando al Regolamento in modo ampio. La verità è che non tutti rispettano il Regolamento,

alcuna difficoltà a mettere ancora più in chiaro le osservazioni, ricordando che la prassi per la redazione del processo verbale non ha mai previsto precisazioni in questo senso, ma, considerata la delicatezza dell'oggetto in termini politici, la Presidenza non ha difficoltà

la maggioranza di centro-sinistra è stato ribadito il sostegno all'azione della Guardia di finanza che, come affermato nell'intervento del senatore Gerardo D'Ambrosio, riveste un ruolo fondamentale per la lotta all'evasione

Quanto al merito, nel ringraziare tutti, mi permetto di esprimere solidarietà alla Presidenza del Senato tutta, e in particolare al presidente Marini, per le stesse ragioni che lei richiamava.

mi appello a lei affinché si utilizzi nella precisazione la prassi più ordinaria, anche perché un dato c'è: alcuni di noi, quando votarono,

Si tratta di una precisazione che ben venga, per l'amor di Dio! Non ci opponiamo rispetto ad un verbale che ritengo corretto, nella forma e nella stesura, nel riportare ciò che ieri è accaduto in Aula. Certo, la volontà della maggioranza nell'esprimere il voto sull'ordine del giorno G11 era quella di

con cui era stato esposto l'intero ordine del giorno G11; poi, per una questione tecnica, è stata scorporata quella parte di gratificazione che si voleva dare alla Guardia di finanza.

non è necessario; passa attraverso la volontà di questa maggioranza, che ha voluto gratificare la Guardia di finanza.

Signor Presidente, l'interpellanza 2-00159, firmata dal sottoscritto e da altri colleghi, parte dalla considerazione che un settore così delicato qual è quello dell'assistenza protesica meritava, da parte dell'attuale Governo, un tipo di considerazione diversa e un'attenzione anche sul piano delle proposte concrete. Ho fatto un po' la storia di quello che abbiamo cercato di fare con il precedente Governo, mettendo in piedi un tavolo tecnico che concluse i lavori nello scorso anno, nel mese di maggio 2006; tra l'altro, lo avevo

che comunque erano interessati, da un punto di vista produttivo, sanitario e professionale, a fare in modo che finalmente si arrivasse a questa rivisitazione e aggiornamento del nomenclatore tariffario, in presenza peraltro di un settore, nel quale lavorano migliaia e migliaia di persone, che aveva chiesto un aggiornamento del nomenclatore per due motivi. era legato a prezzi che risalivano al 1999, peraltro in presenza di un mercato e di un'esigenza di assistenza protesica che è esploso negli ultimi anni soprattutto per quanto

c'era l'esigenza che la parte strettamente sanitaria avesse un ruolo diverso, un ruolo più importante e più serio, e quindi si desse la possibilità a questa parte sanitaria di esprimersi fino in fondo. Facemmo quel lavoro fino a maggio dello scorso anno e facemmo anche

all'epoca già sottosegretario, e il Presidente della Commissione. In quella sede sollecitammo il Ministero della salute a spiegare i motivi per i quali quel nomenclatore non era ancora andato avanti e quindi in qualche modo eravamo sollecitati a fare

Poi, dopo un silenzio che è durato oltre sette mesi, abbiamo appreso da un comunicato stampa che il Ministero della salute aveva messo in piedi un'altra commissione per la revisione dei livelli essenziali di assistenza.

è stata nominata un'ennesima commissione per la revisione del nomenclatore. È vero che i tavoli tecnici ormai abbondano: anche stamattina, in occasione di un incontro con

le dichiarazioni fatte dal Ministro della salute, che abbiamo incontrato più volte, e le dichiarazioni fatte in Commissione sembravano e sembrano andare nell'ottica di chiudere questa partita una volta per tutte. Mi auguro che oggi,

(dai terapisti ai tecnici della riabilitazione, agli ortopedici), ma soprattutto ci diano la possibilità di far sperare tutte quelle persone anziane che oggi si affidano alle

Come è noto, per la modifica e l'aggiornamento di tutti i servizi e prestazioni attualmente inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA), la normativa vigente prevede il coinvolgimento della commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che deve esprimere una valutazione sui fattori scientifici, tecnologici ed economici che depongono a favore delle modifiche, «in relazione alle risorse definite».

appositamente costituito, ha condotto uno specifico approfondimento che ha portato all'elaborazione di una proposta, approvata nella seduta del 18 ottobre 2006. Tale proposta è stata formulata sulla base di una attenta ricognizione delle relazioni tecnico-scientifiche e professionali elaborate nel tempo da tutti i principali "attori" del settore dell'assistenza riabilitativa e protesica, nonché di una collazione dei documenti propositivi acquisiti e delle segnalazioni fin qui prodotte da enti e associazioni a tutela della disabilità, e dalla valutazione dei numerosi dispositivi che sono stati progressivamente introdotti in commercio e, successivamente, validati con successo nell'uso da parte degli assistiti. Nel corso dei propri lavori, il sottogruppo ha preso in visione anche una proposta precedentemente formulata da un gruppo di lavoro sull'assistenza protesica costituito nell'ambito del Ministero della salute nel corso della precedente legislatura corso della precedente legislatura e ha ritenuto opportuno confrontarsi con i suoi autori. A seguito di questo confronto, il sottogruppo, sulla base di approfondite considerazioni, ha ritenuto di poter utilizzare solo parzialmente alcuni contenuti della proposta. Dal momento che lo schema di revisione elaborato dal "Tavolo tecnico per l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario delle protesi", cui fa espresso riferimento l'interpellanza in esame, riproduce la proposta elaborata dal gruppo di lavoro ministeriale, già sottoposta con esito negativo alla Commissione LEA, non è stato possibile dare seguito a tale schema, se non recependone alcuni contenuti marginali. Tale proposta di revisione, dopo il confronto con i principali "attori" del sistema (Regioni, operatori sanitari, operatori economici, utenti, eccetera), costituirà la base per la modifica della disciplina dell'assistenza protesica, con il fine di realizzare l'obiettivo di garantire la prevenzione ed il trattamento della disabilità ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini disabili. La proposta della Commissione nazionale LEA è stata presentata alle categorie sociali, professionali ed economiche direttamente interessate al fine di raccogliere e, nel caso, recepire ulteriori proposte migliorative. Superata tale fase, detta proposta sarà presentata alla Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della procedura di revisione complessiva dei livelli essenziali di assistenza. L'interpellanza in esame fa espresso riferimento ai comunicati stampa dello scorso mese di marzo, con cui è stato segnalato che il ministro della salute Livia Turco ha inteso sollecitare la Commissione nazionale LEA a predisporre la revisione del Nomenclatore prevedendo la disponibilità di sistemi di comunicazione ausiliari di tecnologia più avanzata, recentemente introdotti sul mercato, rispetto a quelli meno sofisticati contemplati nel decreto ministeriale n. 332 del 1999. Si precisa, altresì, che la Commissione su salute e disabilità, recentemente istituita dal ministro Livia Turco per dare voce alle precipue esigenze dei cittadini, è composta da rappresentanti delle principali associazioni ed enti a tutela delle persone con disabilità ed ha il compito di proporre ed elaborare iniziative volte al pieno recupero dell'autonomia ed alla maggiore integrazione sociale, scolastica e lavorativa di queste persone. Questa Commissione ha un ruolo specifico nella definizione del nuovo Nomenclatore delle protesi, dei presidi e degli ausili sanitari, con particolare riguardo alle modalità della sua revisione, al fine di garantire che vengano sempre inseriti in esso con tempestività i prodotti più innovativi. Considerata la presenza, in detta Commissione, della rappresentanza delle associazioni ed enti che si occupano di queste problematiche, il ministro Livia Turco ha ritenuto di coinvolgerla anche nella valutazione della proposta elaborata dalla Commissione nazionale È opportuno segnalare, in particolare, che tra le linee progettuali riguardanti gli "obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale 2007", figura quella relativa alla "facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie". A tal riguardo, si ritiene di vincolare una quota di dieci milioni di euro da ripartire fra le Regioni, al fine di consentire a detti enti di dotare con moderni sistemi di comunicazione un primo "*target*" di pazienti, tra quelli con fonazione di grado 2 (sostanziale perdita della parola), e con motilità di grado 4 (tetraparesi).

prevista una serie di meccanismi di rivisitazione, di revisione delle protesi e dei prezzi che prescindono dalla realtà. Probabilmente chi ha scritto questa risposta alla mia interpellanza, o chi

il fatto che qualcuno voglia tener conto delle esigenze produttive di qualche mondo che, probabilmente, spinge la porta del Ministero della salute perché non è stato rappresentato o di qualche sanitario che non può svolgere alcuna funzione e quindi è da mettere dentro la Commissione.

al membro del Governo, il sottosegretario Gaglione - faccia in modo tale che questo meccanismo celebri, in tempi brevi, la conclusione di questo processo.

proprio oggi, da questa interpellanza e da questa risposta del sottoscritto, possa trovare il modo per chiudere un'operazione seria, che vada a vantaggio esclusivo dei cittadini.

Presidente, l'atto parlamentare in esame ripercorre la complessa vicenda della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Per altro, nonostante la progressiva evoluzione della contrattazione collettiva e la definitiva collocazione dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute nel comparto di contrattazione del personale dirigenziale dell'area 1, non sembrano superati i limiti segnalati dal Consiglio di Stato. Questo parere concerne l'eventuale inserimento nel ruolo unico di dirigenza del personale della sanità appartenente al primo livello dirigenziale ed in piena sintonia con i rilievi formulati anche dalla Corte dei conti ed esclude che il personale in argomento abbia titolo ad essere inserito nel ruolo unico. Infatti, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nella sua originale formulazione, aveva articolato la dirigenza del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale in due livelli, attribuendo al personale medico delle alte professionalità sanitarie di primo livello funzioni di supporto, collaborazione e corresponsabilità, nel rispetto delle direttive del responsabile della struttura di appartenenza, mentre al personale del secondo livello sono state attribuite funzioni di direzione ed organizzazione.

Per il Consiglio di Stato, quindi, le disposizioni normative e quelle del contratto integrativo del personale in questione «si limitano ad inquadrare il personale (...) nei due livelli in cui si articola la dirigenza del Servizio sanitario nazionale». Come poc'anzi ricordato, anche la Corte dei conti si è più volte espressa in merito alla questione. È opportuno precisare, inoltre, che non vi è stato, per i dirigenti sanitari di prima fascia (ex I livello), a differenza dei dirigenti sanitari di seconda fascia (ex II livello), l'accesso alla dirigenza dello Stato mediante la procedura concorsuale prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né può, d'altro canto, ritenersi che il personale in questione ha beneficiato di meccanismi di accesso automatico e generalizzato a tale dirigenza. Il Ministero della salute, avendo, al pari del personale coinvolto, un interesse diretto alla rapida soluzione della problematica, ha condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, un percorso che, attraverso l'adozione del decreto interministeriale dei ruoli dei dirigenti del Ministero della salute, potesse dare una collocazione certa ai dirigenti delle professionalità sanitarie, anche in applicazione delle norme programmatiche contenute nell'articolo 5 dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005. Conformemente alle motivazioni contenute in questa decisione e, in particolare, con riferimento alla consapevolezza che, come dalla stessa Corte rilevato, l'autonomia collettiva non può invadere campi riservati alla legge, come quello della disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, il Ministero della salute si è attivato per riproporre un nuovo decreto interministeriale, contenente le formule di cautela indispensabili per ottenere l'apposizione del visto da parte della Corte dei conti. Un tale provvedimento sembra lo strumento più adatto per dare l'assetto definitivo alla materia, mediante l'inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, perché non appare erroneo individuare proprio in un decreto, come richiede la norma programmatica contenuta nei contratti collettivi vigenti, la definitiva collocazione dei dirigenti sanitari ex I livello nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute. Al riguardo, si segnala che è intendimento dell'Amministrazione inserire detta disciplina del Consiglio dei ministri (da sottoporre all'esame delle organizzazioni sindacali) che, sviluppato congiuntamente al procedimento di adozione del decreto istitutivo dei ruoli, possa consentire di giungere finalmente ad una gestione efficiente ed efficace delle posizioni dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero, oggi resa difficoltosa dalla situazione di incertezza giuridica complessiva. L'attuale quadro normativo determina l'impossibilità giuridica di conferire, ai dirigenti ex I livello, incarichi di seconda fascia. Occorre precisare che, alla luce del ruolo sempre più importante che il Ministero della salute svolge nel sistema sanitario nazionale, appare inequivocabilmente esclusa l'esistenza di un qualsivoglia pregiudizio nei confronti delle professionalità sanitarie in servizio: questa Amministrazione, pur in un'ottica di massima garanzia di parità di trattamento e di opportunità rivolte a tutto il personale ministeriale, si rivolge con particolare sensibilità a questa peculiare peculiare categoria di personale, senza pregiudicare gli interessi e le prerogative dei dirigenti sanitari ex II livello (medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi, psicologi dirigenti di seconda fascia). Del resto, è evidente il rilievo che le professionalità sanitarie rivestono all'interno del Ministero, ove solo si consideri che a capo di tre dei quattro dipartimenti di questa Amministrazione vi sono un dirigente medico, un dirigente veterinario e un dirigente chimico.

partiva da un presupposto recente, cioè dal fatto che, nel dicembre scorso, è stato sottoscritto a livello politico un protocollo d'intesa che riguardava per la prima volta anche i dirigenti delle professionalità sanitarie e che nel gennaio 2007 c'è stata una piattaforma di contratto collettivo integrativo, concordato con le organizzazioni sindacali,

Sottosegretario - ho preso appunti - si starebbe esaminando la possibilità di un nuovo provvedimento, di un decreto che dovrebbe riconoscere tale attività professionale da parte della dirigenza sanitaria e si sta prevedendo

Infine, ho ascoltato il sottosegretario Gaglione, quando diceva che è escluso il pregiudizio nei confronti della dirigenza medico-sanitaria, quindi vi è un riconoscimento, appunto della dirigenza medico-sanitaria.

concernente il cosiddetto piano di rientro per il contenimento della spesa sanitaria e il perseguimento dell'equilibrio economico. Questo piano di rientro prevede la produzione sistematica di un'informazione contabile precisa e dettagliata del sistema sanitario; la realizzazione della contabilità analitica per centri di costo e il controllo di gestione; il completamento della trasformazione in aziende dei policlinici universitari pubblici; l'adozione dei provvedimenti che razionalizzino la rete ospedaliera, la spesa farmaceutica, la spesa per l'acquisto di beni e servizi, e la spesa per il personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La gestione della rete ospedaliera assistenziale rientra nell'autonomia regionale, così come confermato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, L'ospedale «Nuovo Regina Margherita» dispone di 130 posti letto, di cui 47 in regime di *day hospital*; la Regione Lazio ha comunicato che la riconversione dell'ospedale in questione in presidio territoriale di prossimità prevede investimenti in termini strutturali ed organizzativi. Tutte le attività saranno fortemente integrate con l'assistenza territoriale (medici di famiglia, assistenza domiciliare) e con i servizi sociali. Una ulteriore caratterizzazione del presidio è quella relativa alla costituzione in esso di un Centro per la formazione grazie alla realizzazione di aule didattiche e di una sala convegni. All'interno del presidio è prevista anche la realizzazione di un asilo nido per i dipendenti. In riferimento alla situazione edilizia, l'intervento di riorganizzazione prevede che nella porzione di fabbricato prospiciente Viale Morosini e Viale Trastevere e negli spazi retrostanti vengano concentrati gli ambulatori specialistici, e *day-surgery* e la riabilitazione, dal piano rialzato al piano terzo; la continuità assistenziale, al piano terreno; la diagnostica di immagini, nel piano terreno e nel seminterrato; la direzione sanitaria ed amministrativa. Al piano terreno degli altri fabbricati del complesso saranno collocati: le attività ambulatoriali; i servizi di farmacia e il laboratorio analisi; i servizi generali quali cucina, mensa, bar, banca, spogliatoi, alloggi, depositi, sala riunioni con annesso spazio di gestione; i servizi tecnici di supporto. Negli spazi al piano primo che dall'ingresso di Via Roma Libera girano intorno al quadriportico medievale troveranno collocazione le attività di ricovero "H24" ed in particolare: il servizio psichiatrico; l'*hospice* per malati terminali; la residenza sanitaria assistenziale; il centro risvegli per comi prolungati. I locali intorno al quadriportico rinascimentale e gli spazi attualmente utilizzati dal servizio di farmacia (e in parte da archivi e depositi) sono destinati alle attività di formazione di base e aggiornamento professionale e all'attività convegnistica, con il recupero della sala dello Stenditoio. Gli spazi adiacenti all'ingresso al giardino interno di San Cosimato, attualmente occupati dal *day*-*hospital* pediatrico, sono destinati alla realizzazione del citato asilo nido per il personale ospedaliero, da gestire in collaborazione con il Comune. E' previsto, inoltre, l'abbattimento di alcune superfetazioni al piano terreno e al primo piano, con il recupero dell'immobile dal punto di vista architettonico ed artistico. I giardini del quadriportico rinascimentale e di San Cosimato sono destinati anche ad attività assistenziale e riabilitativa specifica di tipo geriatrico e psichiatrico.

il programmino che le hanno dato da leggere è completamento avulso dalla realtà territoriale di Trastevere e di un ospedale che ha 130 posti letto e che vive e opera da tanti anni al centro di un quartiere popoloso popoloso e popolare come questo. La cancellazione di un ospedale non vuol dire la risistemazione del giardino per la riabilitazione, tutt'altro. La cancellazione di un ospedale vuol dire la presa di posizione unitaria del I Municipio contro tale cancellazione. C'è stata un'assemblea, cui ha partecipato l'assessore alla sanità Battaglia, dove tutti gli operatori si sono dichiarati contrari

all'assemblea c'erano esponenti della CGIL, dei DS, di Alleanza Nazionale, di diverse forze politiche e di diverse forze sindacali e tutti hanno detto no alla chiusura), ci mobiliteremo questa decisione. Mi dispiace per la sua risposta, ma è al di fuori da una realtà territoriale necessaria.

il Presidente della Regione Lazio, concernente il cosiddetto piano di rientro per il contenimento della spesa sanitaria e il perseguimento dell'equilibrio economico. Il piano di rientro siglato dall'attuale amministrazione è finalizzato a colmare il consistente disavanzo, che grava sulla Regione e che la precedente amministrazione non aveva compiutamente rilevato e dichiarato: si ritiene pertanto opportuno mettere a disposizione della signoria vostra copia del piano di rientro, nelle cui premesse è illustrato con precisione il quadro regionale di riferimento, insieme con le problematiche di carattere economico-sanitario ad esso connesse, che costituiscono la premessa della razionalizzazione organizzativa attualmente in corso nella Regione. Secondo il piano di rientro uno degli obiettivi indicati per la gestione dei costi è il rispetto degli *standard* nazionali relativi al numero dei posti letto ospedalieri. Tale obiettivo può essere realizzato secondo le seguenti modalità: riconversione e chiusura di ospedali per acuti e cliniche di piccole dimensioni con bassi volumi di attività, o a prevalente attività riabilitativa, in poliambulatori, RSA, presidi territoriali di prossimità o *hospice* per il raggiungimento dello *standard* di 3,5 posti letto per mille abitanti; riconversione e chiusura di reparti per lungodegenza e riabilitazione per il raggiungimento dello *standard* di un posto letto per mille abitanti rappresentati nell'atto parlamentare non può non essere precisato che la gestione della rete ospedaliera assistenziale rientra nell'autonomia regionale, così come confermato della parte seconda della Costituzione». La Regione Lazio ha comunicato che l'allocazione degli ospedali romani non è adeguata alla attuale espansione urbanistica, rendendo così necessaria la presenza di nuovi ospedali nelle aree densamente popolate e la riduzione, ove possibile, degli ospedali esistenti. In particolare, relativamente al Presidio Forlanini, la legge regionale del 28 dicembre 2006, prevede all'articolo 26 che, al fine di razionalizzare e valorizzare il patrimonio regionale esistente, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi un piano di riorganizzazione del patrimonio adibito a sede istituzionale. Tale piano dovrà contenere uno studio di fattibilità per verificare la «possibilità di valorizzare l'ospedale Forlanini come sede delle strutture istituzionali e del Consiglio regionale del Lazio». Lo stesso articolo stabilisce uno stanziamento di 20 milioni di euro «per opere di ristrutturazione finalizzate al trasferimento presso l'Ospedale S. Camillo, delle strutture operanti nel presidio Forlanini». L'Assessore alla Salute ha precisato che i servizi attualmente svolti presso l'Ospedale Forlanini, e ricompresi nei due dipartimenti «Malattie polmonari» e «Neuroscienze» verranno interamente trasferiti presso l'ospedale San Camillo all'interno dei padiglioni denominati «Lancisi» e «Nuovo Traumatologico». Tale trasferimento potrà concretizzarsi entro l'anno 2008, al termine dei processi di ristrutturazione e ammodernamento in corso presso l'ospedale San Camillo. Il trasferimento non comporterà alcuna diminuzione del livello di di attività assistenziale e garantirà comunque la salvaguardia del patrimonio professionale e umano del Forlanini. La struttura attuale del Forlanini verrà destinata ad attività non sanitaria e recuperata come patrimonio immobiliare disponibile per i servizi regionali. Per quanto di propria competenza, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha precisato che il complesso ospedaliero in questione non risulta sottoposto a specifico provvedimento di tutela, emesso ai sensi del Decreto Legislativo 22 l'immobile è sottoposto alla disciplina normativa del decreto legislativo n. 42 del 2004 fino a quando non venga verificato l'eventuale peculiare interesse culturale, a cura dei competenti organi del Dicastero ora

per due motivi. In primo luogo, perché qualche giorno fa con una sentenza del Consiglio di Stato il direttore generale dell'azienda San Camillo-Forlanini è decaduto ed è rientrato il direttore generale che era stato allontanato non per motivi tecnici, ma politici. Dico questo perché, essendo stato presidente dell'Agenzia di sanità pubblica, conosco i dati operativi del sistema sanitario regionale e so perfettamente che il dottor Domenico Alessio, che ha vinto il ricorso e che dovrà essere reinsediato alla guida del San del San Camillo-Forlanini, è contrario, per esempio, alla vendita del Forlanini, mentre invece era favorevole l'attuale direttore generale che viene a decadere con la sentenza del provvedimento del Consiglio di Stato. La richiamo su una questione, gentile Sottosegretario; qualche giorno fa, il dottor Macchitella, che è il direttore generale che ha messo in piedi l'operazione per vendere il Forlanini, ha acquistato per il Forlanini - lui che dice di fare i trasferimenti - una nuova TAC perché la vecchia non funzionava. Ci siamo informati perché quella vecchia non funzionava: aveva un piccolo tubo guasto

le voglio ricordare, per esempio, che il vice presidente della Camera dei deputati, onorevole Leoni, è tra i firmatari della difesa dell'ospedale Forlanini, insieme a registi parlo di registi della cinematografia italiana - attori e personaggi della cultura: c'è un elenco di 160 personaggi della cultura, del cinema, del giornalismo e della politica che hanno firmato un appello alla Regione un appello alla Regione affinché il Forlanini non venga venduto, perché noi lo trasformiamo da struttura ospedaliera in struttura amministrativa. Il direttore generale di quell'azienda è stato denunciato in Consiglio regionale. Si tratta di colui che ha preparato la vendita del Forlanini e che ha addirittura

di portavoce, con lo stipendio adeguato. Dunque, si continua a fare sperpero in quell'azienda ospedaliera e intanto si taglia e si chiude una struttura

senza pensare, ad esempio, che nei giorni passati vi è già stato trasferito il centro trapianti del professor Santoro e quindi non ci sono gli spazi per permettere ad una struttura di livello come quella che opera all'interno del Forlanini di essere trasferita nell'ospedale San Camillo. Ci sono delle incongruenze veramente gravi che riguardano il piano di rientro. Inoltre, abbiamo appreso anche un'altra cosa, e cioè che in questi giorni proprio l'assessore alla sanità della regione Lazio è stato messo sotto controllo perché è stato nominato l'onorevole l'onorevole Cosentino, già assessore alla sanità della regione Lazio fino al 2000, come responsabile della sanità e dunque l'assessore è stato messo un po' all'angolo. Ci auguriamo che, nei prossimi giorni, con il cambio di deleghe all'interno della Regione Lazio, arrivi un assessore, sempre dell'Ulivo, che comprenda che una struttura importante come l'ospedale Forlanini non può essere svenduta per metterci uffici amministrativi, anche se della stessa

Signor Presidente, senatore Domenico Gramazio, rispondo alla sua giusta preoccupazione per un altro ospedale storico

(IFO) di Roma ha inteso sottolineare che le affermazioni riportate, relative al fatto che «il San Gallicano rischia di scomparire», sono previsioni destituite di qualsiasi fondamento sia formale sia sostanziale, come in effetti verificabile sulla base del complesso degli atti deliberativi e delle decisioni fino ad oggi adottate dalla Direzione generale degli IFO. In particolare, lo stesso direttore generale ha dichiarato che non vi è alcun piano di «scomparsa» dello storico ospedale San Gallicano dalla città di Roma, stanti le univoche ed omogenee decisioni delle amministrazioni susseguitesi in precedenza presso gli IFO, che prevedevano appunto l'allocazione di entrambi gli Istituti (Regina Elena e San Gallicano) nel nuovo complesso ospedaliero IFO di Mostacciano. Non vi è alcuna intenzione di «alienare» la struttura del San Gallicano, in quanto la stessa, facente parte integrante del patrimonio degli IFO, è stata affidata, in gran parte e dal 2002, in concessione alla Comunità di S. Egidio con apposito accordo intervenuto con la Regione Lazio e con avallo del Ministro della Salute *pro tempore.*

come operatore in quella struttura da circa 32 anni e ne è diventato da poco il direttore scientifico. È un dermatologo di fama nazionale ed internazionale:

che l'IFO sta dando alla struttura del San Gallicano, perché sono terrorizzato dalle dichiarazioni rese dal professor Di Carlo in Commissione

la sua conoscenza e anche il suo peso all'interno del Ministero della salute, per guardare con attenzione ad una struttura che è orgoglio del servizio sanitario pubblico italiano.

previdenza sociale*. Signor Presidente, in riferimento all'interrogazione presentata, relativa alla posizione dei lavoratori delle cooperative di utilità sociale convenzionate con il Comune di Napoli, passerei prioritariamente ad illustrare quanto comunicato dalla prefettura di Napoli, per il tramite del Ministero dell'interno, che ha ripercorso brevemente le vicende relative alle cooperative in questione. Le Cooperative di lavoro impegnate in lavori socialmente utili per conto dell'amministrazione provinciale e del Comune di Napoli, sono state costituite a far data dal 1980, per progetti di pulizia ed in seguito anche per progetti concernenti la toponomastica, manutenzione patrimoniale, guardiania, verde pubblico e Gli enti sopracitati hanno avviato al lavoro, con diversi provvedimenti deliberativi, circa 4.200 unità inserite in 36 cooperative, di cui 11 convenzionate con la Provincia di Napoli e 25 con il Comune di Napoli. A seguito dell'attivazione delle procedure di liquidazione per 3 cooperative, il numero delle stesse operanti per il Comune di Napoli è passato a 22, con conseguente riduzione dei soci a 3.090 unità, di cui 1.747 impegnate per il Comune di Napoli e 1.343 per la Provincia. L'attività dei commissari governativi viene coordinata, controllata e coadiuvata da un commissario coordinatore del Ministero dell'interno, mentre i servizi amministrativo-contabili vengono effettuati in via esclusiva dal centro unico servizi che ha una contabilità autonoma e le cui risultanze vengono inviate alle autorità di controllo e agli uffici finanziari. La citate cooperative mantengono la veste di società private, ancorché siano contrattualmente impegnate con enti pubblici per lo svolgimento di alcuni compiti, peraltro di interesse sociale, in ragione dei quali ricevono corrispettivi direttamente dagli enti locali, previa presentazione di fatture per i servizi svolti. Queste, infatti, non ricevono direttamente i finanziamenti statali di cui invece sono beneficiari soltanto gli Enti locali interessati appunto alle società cooperative che sono legate con contratto di diritto privato. Attualmente le cooperative convenzionate con il Comune risultano essere 12, mentre per la Provincia 11. Con riferimento a questi lavoratori, come ricordato dal senatore Russo Spena, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997, recante contributi per spese pubbliche nei Comuni di Napoli e Palermo. In proposito, il Ministero dell'interno ha reso noto che la Giunta del Comune di Napoli ha operato la ripartizione del ricordato finanziamento per l'area del napoletano, il Comune ha sottoscritto con i rappresentanti delle cooperative ancora in esercizio un'apposita convenzione che regola i reciproci rapporti ed individua le aree di attività alle quali sono destinate le prestazioni dei soci, ovvero: area 1, pronto intervento di pulizia, piccola manutenzione strutture comunali; area 2, vigilanza, sorveglianza strutture e aree di pertinenza comunale; area 3, socio-culturale educativa; area 4, organizzativa e amministrativa. Il Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha reso noto, in merito alle attività del cosiddetto "Tavolo per Napoli" recentemente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del quale è coordinatore, e del quale è coordinatore, che tale organismo consiste in una unità speciale di concertazione per lo sviluppo di Napoli e della sua area, strumento di coordinamento amministrativo tra il sistema degli enti locali e il Governo centrale, nonché in una unità tecnica che riunisce i rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte. In particolare, il Dipartimento sopra menzionato ha comunicato quanto segue. Ai lavori della suddetta unità tecnica partecipano, per il Comune di Napoli, il segretario generale, quale rappresentante permanente dell'amministrazione comunale, nonché l'assessore con deleghe al lavoro, alla cultura e ai grandi eventi. Finora la sessione di lavoro dei suddetti organismi ha affrontato i temi connessi all'insediamento di nuove imprese ICT nell'area napoletana, alla realizzazione dell'aeroporto di Grazzanise, al completamento della rete metropolitana comunale e regionale, ai risultati del piano sicurezza, alla candidatura di Napoli ad ospitare il *forum* delle culture UNESCO del 2013. Con riferimento specifico a quanto aggetto dell'interrogazione in esame, il richiamato Dipartimento ha fatto presente che, nelle sedi sopra richiamate è attualmente in corso un positivo confronto volto ad individuare nuove politiche per l'assistenza e la solidarietà, idonee a superare i limiti delle esperienze finora realizzate, consistenti essenzialmente nella previsione di sussidi minimi di inserimento e di iniziative per la formazione. Su tali basi, l'unità speciale per Napoli viene considerata dalla Presidenza del Consiglio quale sede idonea ed affrontare ed analizzare, in termini sia politici che tecnici e tenendo adeguatamente conto delle richieste dell'amministrazione locale direttamente coinvolta, i temi relativi alla posizione dei lavoratori delle cooperative di utilità sociale convenzionate con il Comune dì Napoli.

Sono, inoltre, in grado di informare che è in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* la circolare con la quale sono indicate le modalità di attuazione della norma di legge (articolo 1, comma della legge finanziaria 2007) che prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'erogazione di incentivi a carico del Fondo per l'occupazione in caso di assunzione di soggetti già impegnati in attività socialmente utili presso i Comuni medesimi. L'incentivo previsto per tali assunzioni, che dovranno avvenire nei corso dall'anno 2007, è pari a 9.296,22 euro annui par ogni contratto dì lavoro stipulato a tempo pieno o parziale e comunque indeterminato. Le assunzioni interessano Comuni che presentino vuoti nella relative dotazioni organiche del personale ed interessano le qualifiche lavorative per le quali non è richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuoia dell'obbligo. Il numero massimo complessivo dalle assunzioni è pari a 2.450 di queste, il 60 per cento sarà assegnato ai Comuni che appartengono alle Regioni ammissibili nell'anno 2007 all'obiettivo 1 della Commissione europea nelle quali le percentuali di lavoratori socialmente utili impegnati nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Infine, sottolineo che nei prossimi giorni, per quanto riguarda il Ministero e per la delega conferitami dal Ministro del lavoro, ho già in programma un incontro con gli amministratori locali relativamente alla situazione generale che riguarda quel territorio per quanto attiene ai lavoratori socialmente utili per confrontare ipotesi che anche l'Amministrazione comunale di Napoli ha cominciato ad avanzare, perché quell'incontro diventa importante all'interno di un quadro generale e di una programmazione che il Ministero sta predisponendo in relazione ai 21.000 lavoratori socialmente utili che a livello nazionale

Tuttavia, non sono soddisfatto, non della sua risposta, ma della mancanza di una proposta di soluzione che per la verità individuo forse anche in un limite degli enti locali (Comuni, Provincia, la stessa Regione), come in parte si evince anche dalla cronistoria della complicata vicenda occupazionale che riguarda gli ultimi trent'anni a Napoli. Per dirla con una battuta, è evidente che abbiamo vari problemi: quello dei lavoratori socialmente utili, quello di questi lavoratori delle cooperative di salario sociale, di reddito di cittadinanza; tuttavia, converrebbe avere una strategia globale con punti specifici e precisi. Chiedo, in particolare, una proposta specifica che riguardi questi lavoratori precari delle cooperative di utilità sociale che da vent'anni, sulla base della legge n. 452 del 1987 e successive modificazioni, ogni anno in finanziaria ricevono un finanziamento (quest'anno di 100 milioni, che per la verità riguarda anche in parte Palermo), cooperative

e dopo la lotta del movimento disoccupati a metà degli anni '70, da una parte, e, dall'altra, dalla sensibilità dell'allora cardinale della Chiesa napoletana e del sindaco *pro tempore* Maurizio Valenzi, che vollero porsi il problema del reinserimento sociale degli ex detenuti, e sulla base di un bando, signora Sottosegretario, promosso dall'allora Ministro del lavoro, onorevole Foschi. Il punto è che non servono soldi - ecco la forza della proposta che io tento di avanzare - per la stabilizzazione di questi precari, a differenza dell'altro problema che pure lei opportunamente segnalava, quello della stabilizzazione degli LSU; servono solo norme e decisioni politiche. Lavoratori che svolgono - l'ha detto lei - un ruolo insostituibile nel Comune di Napoli e nella Provincia, con opportune convenzioni (pulizie, piccole manutenzioni, vigilanza, sorveglianza, settore socio-culturale),

un'iniziativa tesa a superare i commissari, ad assumere questi lavoratori a parità di spesa a ruolo speciale e magari lavorare per un prepensionamento volontario; sono convinto che alla fine ci sarebbe un risparmio e una maggiore efficienza - è questo che chiedevo nell'emendamento - al fine di permettere piena efficienza della pubblica amministrazione. Mi avvio a concludere, ringraziandola molto per i dati che ha fornito al monitoraggio. C'è un nesso, ha ragione lei, con quel tavolo per Napoli, l'unità speciale per lo sviluppo dell'area metropolitana, coordinato dalla Presidenza del Consiglio, anche qui per dare per dare più servizi ai cittadini; c'è una positiva iniziativa del Comune e della Regione per una agenzia strumentale che assorba tutti i lavoratori precari e un positivo confronto in atto. Tuttavia, signora Sottosegretaria, mi soffermerei di più sulla proposta specifica che riguarda questi lavoratori delle cooperative di utilità sociale